Grazie Signori senatori, il 2 agosto del 1980 fu inferta al nostro Paese una ferita insanabile. Alle ore 10,25 di quel sabato 85 innocenti persero la vita e oltre 200 tra tra uomini, donne e bambini rimasero feriti. Se alla stazione di Bologna tuttora c'è l'orologio fermo per sempre a quel drammatico momento, a ricordarci fin dove possono arrivare l'odio e l'orrore, le istituzioni hanno il dovere di fare in modo che il tempo non sia passato invano e non solo per impedire il ripetersi di gesti così folli, ma anche per lenire il dolore con tutto ciò che si ha a disposizione. Non ci possono essere zone d'ombra, a partire dalla ricerca di tutti i colpevoli e di tutte le connivenze. Questa non è, non può e non deve essere l'occasione per polemiche di alcun tipo. Oggi è il giorno in cui dobbiamo onorare le vittime, le loro storie e le loro vite e ricordare a noi stessi come il Paese sia riuscito, anche dopo quell'infausto giorno, a rialzarsi e a ricostruire le ragioni del nostro stare insieme, i valori della nostra comunità nazionale, i principi alla base del nostro Stato di diritto. Abbiamo ogni giorno il dovere di coltivare e tramandare la memoria di quanto accaduto, di come il terrorismo abbia cambiato per sempre la storia italiana dello scorso secolo e di come sia stato sconfitto a tutti i livelli. L'Italia non si arrese e seppe trovare, in nome della libertà e della democrazia, la forza per costruire un Paese migliore e pacificato. Alle famiglie delle vittime giunga il sentito cordoglio dell'Assemblea del Senato della Repubblica. Invito tutti i colleghi ad osservare un minuto di raccoglimento.

Grazie

L'episodio si inserisce in un quadro in cui troppo spesso è accaduto che ci fosse uno spazio troppo ristretto per le domande e gli interventi, non soltanto dei Gruppi, ma dei singoli senatori. Noi abbiamo sempre collaborato per rendere possibile lo svolgimento di questo importante atto della vita delle Commissioni, ma lamentiamo il fatto che troppo spesso gli spazi siano stati estremamente ristretti, al punto da poter parlare due, tre, a volte cinque minuti per Gruppo: il che pare davvero non sufficiente. Ieri mattina, quando una collega ha chiesto conto di due domande che aveva posto e alle quali il Ministro non ha risposto, c'è stata da parte del Ministro una reazione francamente inappropriata ad un'Aula parlamentare,

lo spirito dell'audizione, che dovrebbe essere una esposizione chiara, senza assalti da parte di nessuno: si vuole sapere dai Ministri, in questo caso da quel Ministro, quali sono le sue linee programmatiche. Ritengo che questo atteggiamento non sia un accettabile. Non si possono offendere i senatori e la dignità del Senato con atti di questo genere. di questo genere. Visto anche il filmato con l'atteggiamento sia del Ministro che del Presidente della Commissione, che ha, come è suo diritto e dovere, richiamato chi, da parte dell'opposizione, il Presidente della Commissione può dire a un senatore di stare zitto, se è previsto dal Regolamento, ma certamente non può dirlo il Ministro. Auspico che ci sia un rapporto di maggiore rispetto nei confronti dei senatori, del Senato, della Commissione, specialmente in un periodo in cui si sente parlare, da esponenti autorevoli di un importantissimo movimento politico, di abolizione del Parlamento e di sorteggio dei parlamentari, che equivale all'abolizione del Parlamento. Dunque, non possiamo

intervengo in risposta all'intervento del senatore Malan. Ieri ho avuto l'onore di presiedere la Commissione agricoltura in occasione della relazione del Ministro sulle linee programmatiche

in maniera esauriente, che ogni qual volta vi sarà un problema, anche su temi specifici, arriverà in Commissione a spiegare quali sono le linee programmatiche del Governo e le possibili soluzioni a eventuali problemi del mondo dell'agricoltura.

sia possibile chiudere qui l'incidente, anche perché dobbiamo occuparci di temi sicuramente ben più importanti. Il mondo dell'agricoltura, lo sappiamo, è in difficoltà. Continuiamo a parlare di agricoltura, che credo sia la questione che più interessa i nostri agricoltori e tutti i cittadini.

di una mia dichiarazione, si è permesso di dire, davanti a tutti i sindaci, che in questo Parlamento noi perdiamo tempo, mentre lui era lì a lavorare, rinunciando alle ferie. Pertanto, parliamo di una persona che - evidentemente - è vocata all'offesa del Parlamento e dei parlamentari.

Ha chiesto di intervenire il Presidente della 1ª Commissione permanente, senatore Borghesi, per riferire sui lavori della Commissione in ordine al disegno di legge n. 717, di conversione in legge del decreto-legge 25 luglio

domani alle ore 9,30.

nella mia Commissione, e, per quel che ho potuto sapere, anche nella Commissione bilancio. Ci siamo trovati di fronte a due riunioni della Commissione completamente improduttive: una volta mancavano i pareri di ammissibilità, poi i pareri di valutazione finanziaria della 5a Commissione. Ci siamo riconvocati. Il presidente Borghese - gliene do atto - ha provveduto ad assolvere al proprio dovere; ci ha fatto avere i pareri di ammissibilità ma, ancora una volta, si siamo trovati privi dei pareri sulla ricaduta finanziaria del provvedimento.

che ci inquieta, perché non ci siamo potuti esprimere come avremmo voluto sugli emendamenti che il nostro Gruppo ha presentato. Riteniamo che questo fenomeno (relazioni tecniche tardive, assenza di risposte) sia qualcosa che va contro il diritto del Parlamento di approfondire i provvedimenti. *(Applausi dal Gruppo PD).* È una situazione particolarmente grave, signor Presidente - me lo lasci dire per altre ragioni che voglio brevemente esporre. La prima che è ci troviamo di fronte alla prima lettura di un provvedimento molto complicato, uno dei più complicati che il Parlamento deve affrontare, come il milleproroghe. Questa Assemblea, questo ramo del Parlamento, lo esamina in prima lettura, e probabilmente non avrà un grande approfondimento nell'altro ramo del nostro Parlamento, perché sappiamo che così vanno le cose nel nostro ordinamento. Dato che si tratta della prima lettura, la compressione dei lavori delle Commissioni è particolarmente sconveniente e ci allarma. Dico di più: non abbiamo insistito noi perché questo provvedimento fosse incastrato nel calendario dell'Assemblea in questo momento. È la maggioranza che lo ha fatto, e dovrebbe fare tutto il possibile perché il lavoro in Commissione possa svolgersi ordinatamente. Infine,

dare. Di fronte al primo complesso provvedimento emanato con decreto-legge, allora, ci troviamo dinanzi a un tentativo che va in direzione completamente opposta: probabilmente avremo una maggiore

Presidente, questa valutazione che esprimiamo rispettosamente, ma con estrema fermezza, è di grande forza perché intravediamo una volontà: c'è la sensazione che alla fine a queste contraddizioni si cercherà di porre

l'incapacità di organizzare i lavori e di operare con efficienza da parte della maggioranza e del Governo. Quindi, le chiediamo di vigilare, per quanto in suo potere, affinché questo non avvenga. Capisco la devozione con cui i rappresentanti della maggioranza ascoltano i discorsi sulla democrazia morente e sul Parlamento superato, ma il Parlamento ancora c'è, e finché c'è va rispettato. *(Applausi dal Gruppo PD).* Anche quanto detto dal senatore Malan e dagli altri senatori dovrebbe essere ragione di grande preoccupazione. Capisco il senatore Vallardi. Non si è trovato in una posizione facile, però vorrei dirgli che le difese d'ufficio sono sempre imbarazzanti. *(Applausi della senatrice Malpezzi).* Quando si nutrono di lotta all'evidenza diventano doppiamente imbarazzanti.

e posso garantirle che i nostri predecessori ci hanno fatto aspettare molto tempo, e noi con pazienza abbiamo sempre aspettato. Quindi chiederei gentilmente alle opposizioni di fare il possibile per accettare una richiesta di tempo strettamente necessaria a valutare la portata finanziaria di tutti gli emendamenti. Signor Presidente, mi scuso se interloquisco in questo momento con lei e con l'Assemblea, ma vorrei attribuire anche qualche motivazione e responsabilità rispetto a quanto sta accadendo.

stortura avevo posto rimedio con una proposta di modifica del Regolamento, portata in Aula, che prevedeva che la Commissione bilancio si sarebbe espressa solo sugli emendamenti approvati in Commissione e su quelli portati in Aula.

Grazie alla presentazione di un emendamento del senatore Tonini, allora Presidente della Commissione bilancio, quella

Parliamo di una situazione, signor Presidente, molto grave. Io credo che non si debba permettere ad alcuni colleghi di ricostruire la storia, compresa quella della modifica del Regolamento della quale, a seconda dei momenti e a fasi alterne, ci si prende il merito o meno. se il Presidente Calderoli è responsabile di questo Regolamento, lo ha detto con vanto recentemente in quest'Aula, è responsabile anche di quanto sta succedendo oggi.

di lanciare questo tipo di messaggio. Quando il Parlamento si riunisce e discute su questioni rilevanti mette in evidenza l'incapacità di questo Governo e di questa maggioranza di preparare gli atti *(Applausi dal Gruppo PD)*, mette in difficoltà le Commissioni. Autorevoli colleghi, le Commissioni sono state ferme per ore, per giorni, semplicemente per l'incapacità di preparare adeguatamente gli atti parlamentari. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Credo che la maggioranza abbia solo un modo per affrontare la situazione: da una parte cominciare a lavorare seriamente sui provvedimenti che presenta in Aula e al Paese, e dall'altra semplicemente chiedere scusa a noi e a tutto il Paese per lo spettacolo tremendo di incapacità *e M5S**)*, di ignoranza, di improvvisazione e di superficialità che la Lega e il MoVimento 5 Stelle stanno dando all'Italia.

Stava protestando ed è uscito. ma non capisco niente di quello che dite, perché urlate. Mi pare che il vostro Capogruppo, il senatore Marcucci, abbia espresso il suo dissenso. LAUS *(PD)*. Prima

Prima di sospendere i lavori, vorrei formulare i miei complimenti più vivi al senatore Casini, che è stato eletto Presidente del Gruppo italiano dell'Unione interparlamentare. Presidente Casini, auguri vivissimi.

Signor Presidente, egregio signor Ministro, l'Italia è penultima in Europa nella classifica per tasso di occupazione delle donne, con una differenza tra il tasso di occupazione maschile e quello femminile che sfiora il 20 La drammaticità della situazione italiana è ulteriormente peggiorata dal fatto che, mentre negli altri Paesi europei alcune forme di flessibilità del lavoro (come il *part time*) contribuiscono ad evitare un incremento del tasso di disoccupazione, in Italia invece l'accesso al *part time* è molto limitato, non essendovi alcuna garanzia a livello normativo che favorisca le donne con figli piccoli, con conseguente scelta obbligata di licenziamento. Inoltre l'Italia stenta anche sul numero di donne laureate e sul numero di figli per donna, con percentuali fortemente al di sotto della media europea. Per le donne è sempre più difficile conciliare lavoro e maternità, con conseguente naturale diminuzione del tasso di natalità. Sarebbe pertanto necessario rimuovere tutti gli ostacoli che disincentivano le donne dal cercare un lavoro, distribuendo in maniera più equa l'impegno familiare tra uomo e donna. Purtroppo nel contratto di Governo le donne sono menzionate come gli unici soggetti responsabili del dover conciliare i tempi da dedicare alla famiglia e al lavoro. Infine, molte delle misure introdotte dai precedenti Governi a sostegno delle madri sono in scadenza. Se non verrà rinnovato, scomparirà il cosiddetto *voucher baby sitter* per le donne che decidono di rientrare al lavoro, nonché il congedo di paternità obbligatoria, anch'esso in scadenza a fine 2018. L'interrogante chiede di sapere se da parte del Ministro vi sia consapevolezza della problematica espressa e quali misure intenda adottare per ridurre il divario con gli altri Paesi europei, valorizzando il talento femminile, favorendone l'alta formazione e introducendo nuove e apposite misure a sostegno delle madri che lavorano o, quantomeno, se intenda garantire il rifinanziamento delle misure già introdotte dai precedenti Governi.

un *gender gap* molto marcato e un differenziale tra maschi e femmine in termini di occupazione pari al 19 per cento in media su tutto il territorio nazionale. A livello regionale ci sono molte variazioni e si va da un valore minimo di 10 punti percentuali di differenza in Valle D'Aosta a un valore massimo di 25 punti percentuali in Sicilia. La prima missione di questo Governo è riconoscere adeguate tutele ai lavoratori più deboli, superando forme di precariato e discriminazione. Le donne purtroppo rappresentano ancora una fascia particolarmente vulnerabile nel momento dell'ingresso e della stabile permanenza nel mondo del lavoro. In vista della prossima legge di bilancio, stiamo valutando un quadro di interventi in grado di assicurare risposte efficaci e durature. Stiamo valutando una razionalizzazione e una stabilizzazione di misure di sostegno finanziario alla natalità attualmente previste. Vogliamo investire nelle famiglie italiane e far sentire loro la vicinanza dello Stato in ogni momento in cui ne hanno bisogno. In particolare, stiamo considerando la possibilità d'introdurre una misura forte, di copertura totale del costo per gli asili nido, in modo da favorire la conciliazione famiglia-lavoro. Alla copertura degli oneri si potrà provvedere anche con risorse comunitarie del Fondo sociale europeo, oltre che con una riorganizzazione di diversi contributi, attualmente frammentati. Infine, dal momento che c'è un forte legame tra bassi tassi di occupazione e bassi tassi di scolarizzazione, vogliamo intervenire nel medio periodo su programmi mirati verso donne, giovani madri e donne con bassi tassi di scolarizzazione. Solo il 25 per cento delle donne con una licenza di scuola media lavora, mentre il 75 per cento di donne con una laurea lavora. Agiremo quindi su programmi mirati e sull'accrescimento delle competenze. In questa direzione va anche l'introduzione dello strumento del reddito di cittadinanza. *(Applausi intervenire in replica la senatrice Unterberger, per due minuti. Avrei però una preghiera, colleghi: in Aula non si fanno foto con i cellulari.

che non può lavorare perché non ci sono misure che permettono la conciliazione tra lavoro e famiglia. Purtroppo, come ripeto sempre, nel vostro contratto di Governo si parla delle donne nel capitolo delle misure per la famiglia e quando si parla di misure per la famiglia si parla solo dei compiti delle donne. In futuro, anche gli uomini

in questi primi mesi di Governo - e anche nel suo precedente impegno politico - nei confronti della lotta ai cosiddetti privilegi, cosa sicuramente condivisibile, specialmente a fronte di quanto emerge dalle statistiche - com'è per esempio della Svimez, sul Mezzogiorno, o dell'Istat, sul crescente aumento della povertà in Italia e delle diseguaglianze tra ricchi e poveri e tra Regioni ricche e povere.

regole contributive diverse dagli altri lavoratori perché possono vedersi ugualmente versati i contributi (o addirittura lo stipendio) da enti terzi rispetto al sindacato presso cui prestano effettivamente il proprio lavoro e perché possono, prima di andare in pensione, farsi pagare dalle organizzazioni sindacali incrementi delle proprie pensioni a condizioni molto vantaggiose. I sindacalisti svolgono una funzione assolutamente necessaria nel nostro Paese. Proprio per questo, trattandosi di una funzione necessaria che risponde anche alla vocazione etica di tutelare e rappresentare i lavoratori, dovrebbero avere, come chiunque altro svolge rappresentanza politica, sociale e sindacale, un comportamento che non sia

privilegi. Essi riguardano certamente anche i contributi figurativi, come altre categorie; riguardano il distacco sindacale, soprattutto quando è fatto da enti pubblici - che sono tanti e troppi

traggono beneficio e, inoltre, se intende procedere al ricalcolo delle pensioni anche…

Signor Presidente, ringrazio il senatore interrogante. Innanzitutto tengo a ribadire in quest'Aula che questo Governo, così come è previsto dal contratto di Governo, vuole mettere fine a tutti i privilegi, vitalizi, auto blu e pensioni di privilegio.

chiaramente interverremo. Stiamo già lavorando, in collaborazione con l'INPS, per eliminare le cosiddette pensioni d'oro e le dico che nulla osta, secondo questo Ministero, a metter mano alla pensione dei sindacalisti. La peculiarità dell'ordinamento previdenziale per i sindacalisti consente loro di avere una pensione di privilegio incrementando la retribuzione pensionabile negli ultimi anni di servizio. Il versamento della contribuzione aggiuntiva produce, infatti, un incremento delle quote di pensione calcolate ancora con il sistema retributivo, in quanto risultano agganciate allo stipendio degli ultimi anni di servizio. Peraltro, c'è una notevole disparità di trattamento tra sindacalisti che sono dipendenti pubblici o iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria e sindacalisti che non lo sono. Interverremo in maniera risoluta per impedire che questi privilegi vengano mantenuti. Non sono ammissibili incrementi anomali e cospicui delle retribuzioni dei sindacalisti in un così breve lasso di tempo, senza che nello stesso tempo risultino essersi verificate variazioni negli incarichi di dirigenza sindacale conferiti perché ciò comporta degli sproporzionati privilegi in termini di prestazione pensionistica a danno della finanza pubblica e delle tasse dei cittadini. PRESIDENTE. siamo soddisfatti perché le abbiamo dato questa possibilità di esprimersi finalmente su questo argomento anche in una sede pubblica. Siamo soddisfatti perché ha preso un impegno ufficiale a dare il nulla osta al presidente dell'INPS per eliminare da subito il privilegio più scandaloso:

pronti a giudicarla positivamente con un comunicato, quando lei firmerà il nulla osta. Sono passati due mesi di Governo. Capisco che il tempo è stato dedicato ad altro. Aspettiamo i prossimi giorni per ottenere la notizia e le chiediamo nel contempo, ma lo faremo anche in un altro momento, se come Ministro dello sviluppo economico vorrà dare continuazione anche al provvedimento, non riproposto dal Ministro precedente, in merito ai tetti degli stipendi dei *manager* pubblici, che nel frattempo, in mancanza di un suo provvedimento,

fino al 32 per cento. Il reddito di cittadinanza che volete introdurre a me pare che sia uno strumento abbastanza pericoloso, perché, soprattutto al Sud, potrebbe creare quella sorta di di reddito per cui la persona disoccupata non cerca più di reinserirsi nel mondo del lavoro. Peraltro, laddove si dovesse reinserire, lo farebbe magari svolgendo lavoro in nero, con questo creando un danno alle tante imprese che lavorano rispettando la legge.

le modalità di recupero delle stesse e se e quali misure intende adottare per prevenire eventuali abusi nell'utilizzo di questo strumento.

di questo Governo e la sua istituzione è prevista proprio dal contratto che è stato stipulato tra le due forze politiche di maggioranza. Soprattutto, secondo noi, è una priorità per il Paese. Davanti al continuo impoverimento delle famiglie italiane non si può più restare inermi, né proporre palliativi che non risolvono il problema. C'è bisogno di una vera e propria manovra economica. Secondo l'ISTAT, le famiglie in condizione di grave deprivazione materiale sono oltre l'11 per cento del totale. Il reddito di cittadinanza ha la duplice funzione di togliere le persone dallo stato di povertà in cui vivono e di formare per il lavoro i cittadini che sono disoccupati. Esiste praticamente, in forme diverse, fatta eccezione per l'Italia e per la Grecia, in tutti i Paesi dell'Unione europea. È quindi ora che questa misura a riconoscimento della dignità della persona venga introdotta anche nel nostro Paese. La proposta di legge sul reddito di cittadinanza è pronta e stiamo già lavorando in tal senso in coordinamento con il Ministero dell'economia per gli ultimi dettagli. Avrete modo a breve di discutere tutti i dettagli del reddito di cittadinanza in questo ramo del Parlamento. Dal lato dell'incontro tra domanda e offerta predisporremo una banca dati per la classificazione e l'incrocio dei dati. Il sistema informativo unico verrà alimentato con informazioni elettroniche continue da Ministeri e istituzioni, con la registrazione elettronica di qualifiche e competenze dei lavoratori e con la creazione di un fascicolo personale elettronico. Per contrastare gli abusi, sono previste delle sanzioni pesanti per coloro che dichiarano il falso sulla situazione reddituale o lavorativa e possono così ottenere illegittimamente il reddito. Sono previste sanzioni anche verso i funzionari pubblici responsabili di un'assegnazione illegittima di questo strumento. Allo stesso tempo, i beneficiari devono impegnarsi a trovare lavoro con l'aiuto dei centri per l'impiego riorganizzati e devono rendersi disponibili a lavorare e ad accrescere le loro competenze. Si impegneranno anche in progetti utili alla collettività fino a un massimo di otto ore settimanali e non potranno rifiutare le offerte che saranno loro poste. Oltre ad impegnarsi in una ricerca attiva del lavoro per almeno due ore al giorno, dovranno formarsi, quindi non potranno starsene sul divano.

Signor Ministro, dovrei dirmi soddisfatto della sua risposta, fermo restando che non ha risposto al quesito più importante, ovvero come ritenete di potere avere la somma necessaria per pagare questo reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda le esperienze, posso dirle che, a mia conoscenza, esiste un precedente in Europa di introduzione del reddito di cittadinanza ed è la in Finlandia, dove l'esperimento coinvolgeva 2.000 soggetti. Dopo un anno, l'esperimento è stato interrotto, perché anche in Finlandia chi lo percepiva non cercava altro lavoro. Questo è il problema. Se poi lei mi dice che il lavoro deve essere cercato tramite

riguarda la vicenda dell'aereo di Stato Airbus A340-500, tornata da poco alla ribalta della cronaca politica, la cui situazione contrattuale è stata poco chiara fino a poco tempo fa. Risulta, tra l'altro, che Alitalia sia stata usata o chiamata in causa - quindi è un *dossier* nelle mani dello Sviluppo economico

Ora ci si chiede quale sia l'*iter* procedurale che ha seguito l'attuale Governo per la cessazione degli effetti del rapporto contrattuale; se risultino clausole negoziali che prevedono un'opzione di acquisto del velivolo e - in tal caso - a quale prezzo, e se lo stesso velivolo risulti aver operato una o più tratte o che non abbia quasi del tutto volato; se risulti chi abbia voluto e individuato il velivolo e se vi siano state delle deleghe da parte della Presidenza del Consiglio dell'allora

Con una lettera, io e i ministri Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta abbiamo chiesto formalmente ai commissari Alitalia di risolvere quel contratto, che prevede quattro salatissime voci di spesa: prima di tutto il *leasing*, 81 milioni di euro; poi la manutenzione, 31 milioni di euro; poi l'*handling*, 12 milioni di euro, e l'addestramento piloti, 4 milioni di euro, per un costo complessivo che arriverebbe intorno a 150 milioni di euro in otto anni, con la mancata riconfigurazione interna dell'aeromobile. Si tratta di soldi che non vanno ad Alitalia, il nostro vettore, ma nella quasi totalità a beneficio di Etihad, la proprietaria dell'Airbus A340-500. Stiamo parlando di un quadrimotore *turbofan*, uscito dal mercato nel 2011 e quindi superato e obsoleto; un apparecchio fuori dal tempo, proprio come l'idea stessa di utilizzare questo velivolo per soddisfare esigenze puramente narcisistiche: uno spreco.

Uno spreco multimilionario ai danni dei cittadini italiani. Per noi è una non questione banale, ma di principio. Qualcuno deve rendere conto della totale disinvoltura con cui sono stati usati i soldi pubblici. Qualcuno

di andare fino in fondo a questa storia e svelarne tutti gli opachi dettagli: quanto ci è costato realmente questo velivolo e quali siano stati i veri motivi del suo acquisto. Ricordo che anche la Corte dei conti sta indagando per vederci chiaro.

a sproposito di operazione di propaganda dovrebbe andare a vederlo e poi fare un giro nel mondo reale e constatare - ad esempio - in quali condizioni versano i treni regionali usati ogni giorno da migliaia di pendolari italiani. Allora, se continuate in questo modo, devo interrompere la diretta televisiva. Si farà così. Non ammetto che vi siano offese.

Colleghi, non vorrei arrivare al punto di farvi uscire dall'Aula. Se qualcuno qua dentro vuole offendere, sarò costretta a farlo uscire. Non trovo dignitoso per la politica, le istituzioni e questo Parlamento avere un atteggiamento di siffatto tipo. Ognuno dice quello che vuole, ma le offese non sono ammesse in quest'Assemblea. Non c'è bisogno di offendere

Sono certa che questo Governo non userà più la compagnia nazionale Alitalia per altri fini. Signor Ministro, la ringrazio per la risposta e grazie anche all'opposizione per aver dimostrato che stiamo facendo un ottimo lavoro.

Signor Presidente, dispiace che il ministro Di Maio vada via, perché credo che la domanda dovrebbe in qualche modo interessare anche lui. Ministro Centinaio, lei conosce perfettamente i dati ISTAT relativi al 2017, che confermano, ancora una volta, che il settore primario è tutt'ora fortemente interessato da forme di illegalità nei rapporti di lavoro, con irregolarità rilevate che riguardano il 39 per cento dei rapporti di lavoro dipendente.

Di questi, più di 132.000 sono in condizione di grave vulnerabilità sociale e forte sofferenza occupazionale. Questi numeri, purtroppo, confermano uno scenario simile degli anni precedenti: più di 300.000 lavoratori agricoli, ovvero quasi il 30 per cento del totale, lavorano meno di cinquanta giornate l'anno. È proprio in questo bacino in cui, presumibilmente, si annida il lavoro irregolare e grigio. Il tasso di irregolarità dei rapporti di lavoro in agricoltura è

di civiltà giuridica, di lotta contro le mafie e la criminalità organizzata. Non ritiene, quindi, lei, Ministro, che bisogna andare avanti nell'applicazione della legge, magari mettendo mano alle nuove disposizioni per quanto riguarda anche la parte sul trasporto e il

rilevo in premessa che sulle questioni rappresentate dagli interroganti, il Ministero è coinvolto direttamente in modo particolare per quanto riguarda la Rete del lavoro agricolo di qualità e la relativa cabina di regia, che costituiscono uno dei punti dell'azione di prevenzione del fenomeno del caporalato e del lavoro nero in agricoltura previsto dalla legge n. 199 del 2016. Tale norma si caratterizza per due componenti: una repressiva, che fornisce nuovi strumenti - come la confisca - e inasprisce le pene per chi sfrutta manodopera in stato di bisogno senza più la necessità di dover dimostrare l'uso della violenza come in passato; una preventiva, che mira a valorizzare le imprese in regola attraverso l'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Su questa, il Ministero è fortemente impegnato e intende continuare a promuovere lo sviluppo di tale strumento anche attraverso l'incentivazione delle sezioni territoriali. Con la norma si è esteso l'ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete e l'ambito delle funzioni svolte dalla cabina di regia della Rete stessa, che è presieduta dall'INPS e composta da rappresentanti di sindacati, organizzazioni agricole e istituzioni. Allo stato attuale, sono iscritte alla Rete 4.000 imprese. Ritengo che tale risultato vada rafforzato ancora attraverso un'azione di promozione della Rete e di ulteriore semplificazione dell'accesso per le aziende agricole La Rete del lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni previste dalla norma in parola. Tra le attività a esse attribuite, rientra la promozione di iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali. Ad oggi, grazie all'impulso della nostra amministrazione e del commissario di Governo per emergenza criminalità a Manfredonia, è stata creata una sezione territoriale della Rete a Foggia. Analoga richiesta di costituzione della sezione territoriale è stata avanzata dal prefetto per l'area di San Ferdinando- Rosarno. questione *voucher*, molti fra voi si sono detti favorevoli alla modifica della disciplina vigente relativa alle prestazioni occasionali in agricoltura. Uno dei primi interventi di questo Dicastero si è mosso proprio in tal senso, riconoscendo che si tratta di un'esigenza reale, avvertita da parte tanto degli imprenditori quanto dei lavoratori che svolgono il proprio impiego principalmente in alcuni periodi dell'anno e che oggi non riescono a utilizzare lo strumento messo loro a disposizione, perché non rispondente alle reali necessità. Pensando alla stagionalità del lavoro, i settori che risultano maggiormente coinvolti sono quelli dell'agricoltura e del turismo, e sono proprio questi alla base dell'intervento normativo su cui stiamo lavorando. Sappiamo bene che un'impresa agricola che si trovi a gestire, in un determinato periodo dell'anno, una mole di lavoro particolarmente gravosa ha la necessità temporanea di avvalersi di personale aggiuntivo. Si sta, quindi, lavorando in più direzioni, con lo scopo di superare le criticità sia dei vecchi *voucher* sia degli attuali. Prima di tutto, si vuole facilitare l'individuazione dei lavoratori disponibili; in secondo luogo, si vuole ampliare l'arco temporale in cui si può usufruire della prestazione, visto che, soprattutto in agricoltura, le condizioni meteorologiche potrebbero costringere ad un inevitabile ritardo dell'attività. Inoltre, senatrice, si intende facilitare l'erogazione

*voucher*, che noi riteniamo che l'aver reintrodotto le nuove norme sui *voucher*, in particolare in agricoltura, rappresenti di fatto un grimaldello per mettere in discussione quella legge, e le spiego anche perché: lei sa meglio di me che nel contratto nazionale dell'agricoltura è possibile anche l'assunzione giornaliera. Il *voucher*

Significa ancora una volta che siamo pronti per l'ispezione. Per questo motivo, noi ovviamente ci batteremo contro le nuove norme sui *voucher* e, se lei davvero vuole applicare

noi sappiamo che gli aiuti accoppiati riguardano comparti specifici di produzione agricola e sono mirati a sostenere l'attività. Trovano ragione nella peculiare importanza del settore, dal punto di vista economico, sociale e ambientale, e nel fatto che le aziende che vi operano siano siano sottoposte a particolari difficoltà o a criticità di breve o lungo periodo. Su questo piano si annoverano questi ambiti per i quali esiste un rischio di abbandono, di declino della produzione, con ripercussioni negative sull'equilibrio agroalimentare e socio-economico di aree territoriali importanti. Seguendo queste finalità, il 26 luglio la Conferenza Stato-Regioni ha approvato lo schema di decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo che prevede, per l'anno di domanda 2019, l'incremento del sostegno accoppiato previsto dalla politica agricola comune per le misure relative alla coltivazione della barbabietola da zucchero, del riso e del frumento duro. L'incremento del sostegno accoppiato per la barbabietola, il riso e il frumento duro, come specificato dallo stesso Ministero, è stato deciso per incoraggiare gli agricoltori ad assumere impegni ancora più incisivi in termini di sostenibilità dei processi produttivi, unica strada per differenziare le nostre produzioni italiane. Si trattava di un provvedimento molto atteso dal mondo produttivo e di un segnale concreto e deciso verso gli agricoltori. La filiera saccarifera ha un alto valore strategico per il nostro *made in Italy*, in quanto si tratta di una produzione di zucchero 100 per cento italiana, di qualità e che rispetta ogni regola sociale, ambientale, sicura e stabile nel tempo. Il settore dello zucchero, infatti, è reduce dalla fine delle quote a ottobre 2017 e da un processo di ristrutturazione molto forte. Lo stesso vale anche per il problema relativo alla coltivazione del riso. Il comparto sta attraversando una forte crisi. Noi siamo qui, Ministro, per chiedere se al fine di proseguire la linea intrapresa non ritenga opportuno favorire una concertazione tra tutte le parti interessate che coinvolga anche le Regioni, per trovare soluzioni che portino a un riequilibrio dei mercati e a un'equa valorizzazione a livello europeo delle eccellenze. Poi vorremmo sapere se non ritenga utile magari procedere a una valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione di questo decreto-legge in termini di numero di aziende coinvolte e di benefici economici, e magari anche socio-economici, attesi.

aumento del valore del pagamento accoppiato previsto dalla PAC in favore di barbabietola da zucchero, riso e frumento duro a tutela dei bieticoltori e dei risicoltori è stata approvata dalla Conferenza Stato-Regioni il 26 luglio ultimo scorso. Le progressive quotazioni in calo hanno reso necessario un tempestivo intervento per aumentare la redditività delle colture ed evitare che il protrarsi di situazioni particolarmente sfavorevoli e penalizzanti possa causare danni, anche irreversibili, alle aziende del settore bieticolo-saccarifero nazionale. Tali aspetti sono stati posti in varie occasioni all'attenzione delle istituzioni europee al fine di poter attivare misure mirate e specifiche che possano risultare più incisive per la difesa delle nostre produzioni, troppo spesso inficiate da condizioni sfavorevoli nei mercati europei e internazionali. Oltre a un costante monitoraggio sull'andamento dei mercati relativi alle produzioni che rappresentano il vanto del *made in Italy* agroalimentare, particolare risalto sarà attribuito all'etichettatura e alla rintracciabilità dei prodotti agricoli utilizzati in quanto tali o come ingredienti di prodotti agroalimentari. Peraltro, l'incremento del sostegno accoppiato in favore di barbabietole, riso e grano duro mira anche a incoraggiare gli agricoltori ad assumere impegni ancora più incisivi sulla sostenibilità dei vari processi produttivi, unica strada per differenziare le produzioni italiane di eccellenza e migliorarne la competitività sui mercati. La modifica dei pagamenti accoppiati rappresenta pertanto solo il primo passo nella direzione di valorizzare la produzione agroalimentare nazionale, in quanto molto di più dovrà essere fatto per affrontare le sfide che il prossimo decennio ci pone. Sarà necessario utilizzare con intelligenza e sinergia gli strumenti che la futura PAC ci offrirà, inaugurando una stagione di concertazione e condivisione utile a superare le divisioni del passato, sempre nel rispetto delle prerogative costituzionali delle Regioni in materia di agricoltura

Presidente, approfittiamo per ringraziare il signor Ministro per la chiarezza espositiva, ancorché - come recita anche il contratto di Governo che sta portando avanti questa legislatura - gli agricoltori si muovano in un sistema governato da politiche di settore ormai quasi di competenza esclusiva della Politica agricola comune. Troppo spesso i Governi italiani sono stati remissivi e rinunciatari in Europa rispetto alle vere esigenze del settore agricolo nazionale. È necessaria una nuova presenza del Governo italiano a Bruxelles per riformare la PAC.

che riguardano zootecnia, anche il comparto cerealicolo, l'ortofrutticolo e l'itticoltura. Signor Ministro, le auguro,

del senatore Parrini del 10 e 30 luglio scorso e della senatrice Valente del 30 luglio scorso. Considerate le gravi affermazioni che sono state rese dal Ministro della giustizia all'esito della seduta del Consiglio dei ministri del 24 luglio, durante la quale era stato approvato il cosiddetto decreto mille proroghe, a commento della norma che rinvia l'entrata in vigore della nuova normativa sulle intercettazioni, ella, signor Ministro, aveva mosso in maniera apodittica gravissime accuse verso il PD responsabile - a suo dire - di un comportamento diretto a legare le mani alla polizia giudiziaria e alla magistratura, impedendo altresì il diritto all'informazione, pur avendo la consapevolezza che l'obiettivo era esattamente il contrario. Considerato, altresì, che lei ha affermato più volte che uno dei primari obiettivi del Governo di cui lei fa parte è la lotta alla corruzione, che, data la diffusione, minerebbe alla radice le aspettative legittime dei cittadini onesti, prevaricate dal sistema delle raccomandazioni e della corruzione, salvo poi apprendersi dei suoi rapporti con l'avvocato Lanzalone, che come confermato in più sedi, anche ufficiali dalla stessa sindaca Raggi, era stato da lei segnalato proprio alla Raggi quale consulente su questioni rilevantissime, considerato, altresì, che appare quantomeno risibile il fatto che si debba ricordare al Ministro della giustizia che il suo compito precipuo è tutelare il principio di indipendenza della magistratura da condizionamenti del potere pubblico, si chiede di sapere da lei di quali informazioni il Ministro della giustizia sia in possesso per affermare che ogni volta che qualcuno del PD veniva ascoltato c'era il PD che cercava di tagliare la linea e le comunicazioni, chiarendo altresì sulla base di quale legge dello Stato, con quali modalità e con quali finalità ella abbia ottenuto queste informazioni, doveroso, vista la gravità dei fatti riportati, informarne subito il Parlamento. Si chiede di sapere se non ritenga che le sue affermazioni siano state gravemente lesive delle prerogative e dei compiti della magistratura e della polizia giudiziaria e se, nel suo ruolo di Ministro, si sia attenuto al rispetto dell'applicazione delle leggi vigenti, nonché alla tutela delle prerogative e dei compiti di cui ho testé parlato; se, al fine di tutelare il ruolo istituzionale che ricopre, non ritenga necessario chiarire in tempi brevi la natura dei suoi rapporti con l'avvocato Lanzalone, in relazione ai fatti riportati in premessa e in ragione di quali valutazioni abbia inteso indicarlo alla sindaca Raggi come consulente; se in relazione ai suddetti fatti, a tutela del prestigio e dell'integrità delle istituzioni, lei non ritenga doveroso spiegare se dal giorno in cui lei è stato eletto alla Camera dei deputati a oggi siano intercorsi rapporti di natura professionale o di altro tipo

Signor Presidente, innanzitutto mi sia consentito dire che ricordavo, da parlamentare, che il *question time* fosse uno strumento serio e importante, con cui il Parlamento pungola i Ministri sugli atti presi...

non capisco la protesta, per il semplice fatto che sta parlando di una sua esperienza. Non lo condividete, pazienza. Avanti.

Presidente, chiaramente il Partito Democratico avrà la possibilità di replicare rispetto a ciò su cui non concorda. Dicevo, aventi ad oggetto atti del Governo. Non ricordavo che il *question time* fosse uno strumento per trasformare il Senato in un circolo ricreativo per forze politiche che non hanno niente da fare.

Ministro, la pregherei, però...

Chiedo che vengano allontanati dall'Aula i senatori Rampi e Lucidi; che entrambi i senatori vengano allontanati dall'Aula. Chiedo che si allontanino spontaneamente.

vorrei dirle una cosa, con tutto il rispetto che posso avere nei suoi confronti. Siccome non sono riuscita a dirlo prima, perché mi è stato impedito di parlare per il chiasso che si è verificato in questa sede, io vorrei dire che a nessuno è permesso di usare delle espressioni che possano offendere la dignità di quest'Aula. Lo dico a lei e lo dico a tutti.

Cominciamo dai miei rapporti con l'avvocato Luca Lanzalone, in particolare sul perché non l'avrei presentato alla sindaca Virginia Raggi nella mia qualità, allora, di coordinatore dei Comuni governati dal MoVimento 5 Stelle. Io davvero su questo fatto non ho più niente da aggiungere rispetto a quanto ho già ampiamente detto, e cioè che ho presentato un professionista

il mio. Su questo vi dico che, avendo avuto quattr'ore di tempo, non ho potuto preparare nemmeno un testo scritto, ma ho fatto mente locale: negli ultimi sei anni non ho avuto alcun rapporto professionale

emessa dall'avvocato Luca Lanzalone nei miei confronti o viceversa, e non c'è. Spero che adesso questa faccenda possa ritenersi chiusa. Per quanto riguarda le intercettazioni, invece, non mi viene chiesto conto dell'atto, ma della rassegna stampa sull'atto e, in particolare, della mia seguente dichiarazione:

tra l'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi e il comandante Michele Adinolfi. Vuoi vedere che di nuovo per una coincidenza, pochi giorni dopo, il Governo sentiva l'esigenza di far convocare alla Commissione una seduta notturna, nella quale presentava l'emendamento

l'allora *premier* Matteo Renzi e il padre emerse nel caso Consip, l'allora ministro Andrea Orlando dichiarava pubblicamente che il provvedimento sulle intercettazioni andava approvato in maniera celere, proprio per impedire quel tipo di intercettazioni. A questo punto, ho rilevato nella conferenza stampa che c'è una strana coincidenza tra le varie circostanze e ho fatto una mia valutazione politica, che qui ribadisco e sottoscrivo giustizia*. Detto questo, ho notato che le fonti che vengono prese in considerazione sono articoli di giornale e mie partecipazioni a trasmissioni televisive. Visto che la giustizia è una cosa seria, mi auguro che nei prossimi *question time* potremo affrontare con un grande livello di forte critica

che questa sera parteciperò ad una trasmissione radiofonica alle ore 19,30, che potrebbe essere spunto per il prossimo *question time.* Signor Presidente, non possiamo ovviamente che dirci totalmente insoddisfatti per le mancate risposte del ministro Bonafede,

Non ha detto nulla sulla sentenza dei 49 milioni che non viene applicata, né ha detto alcunché soprattutto sulle dichiarazioni di Salvini rispetto al fatto che si sia trattato di una sentenza politica. Questo spetta a un Ministro della giustizia!

e rilevante. La magistratura appurerà le sue responsabilità. Noi siamo garantisti e lo siamo sempre, perché la doppia morale la lasciamo a voi, che cambiate a seconda di dove state, a seconda se sedete in questi o quei banchi. Non vogliamo dire nulla su questo, però le voglio dire una cosa: un Ministro della giustizia parla innanzitutto delle cose che gli competono e, invece, lei, come Ministro della giustizia, di quello non parla. Però è stato solerte e puntuale quando si è trattato di avanzare segnalazioni e raccomandazioni di qualche suo amico collega, in questo caso l'avvocato Lanzalone.

che sono avvocati, che bisogna conoscere un Ministro amico come lei per arrivare a lavorare in qualche studio. Non bisogna studiare. *(Applausi dal Gruppo PD).* Le chiedo merito, Senatrice, vale anche per lei, quello che ho detto prima al Ministro. Vale anche per lei il rispetto che deve a quest'Aula, anche nelle sue affermazioni.

ultima reprimenda che sinceramente non ho compreso. Signor Presidente, credo che ogni parlamentare abbia il diritto di esprimere i propri giudizi e la replica ha proprio questa funzione: esprimere... PRESIDENTE. Basta che i giudizi siano rispettosi. MARCUCCI *(PD)*. I giudizi sono rispettosi per definizione. Se Se la collega ritiene che il Ministro abbia detto delle cose non vere o non sufficienti rispetto alle domande poste dal Partito Democratico, signor Presidente, abbiamo il diritto di dirlo all'Assemblea e al Paese. PD)*. Oggi credo che abbiamo assistito a un pessimo spettacolo: il ministro Di Maio si è fatto preparare l'interrogazione dalla collega per poter dire e fare la sua banale propaganda. Questa non è una trasmissione televisiva; questa è un'Aula parlamentare e si deve rispondere dicendo la verità con la trasparenza nei confronti del Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Signor Presidente, lei ha il dovere di chiedere ai ministri Di Maio e Bonafede di rispettare il Paese e il Parlamento, di venire qua e rispondere puntualmente. Capisco che il collega capogruppo Patuanelli abbia imbarazzo di fronte a queste verità,

la parola quando abbiamo abbandonato l'Aula di fronte alle offese ripetute e chiaramente volute del ministro Bonafede, un Ministro con delle competenze molto particolari. Ogni Ministro ha delle competenze importantissime, ma quello della giustizia più degli altri.

per avere richiamato il Ministro a questa norma di comportamento. Io vedo con preoccupazione il moltiplicarsi di gesti e di parole che non sono rispettosi del Parlamento e della vita democratica in generale. Per questo bisogna tenerli sotto controllo, non ritenerli accettabili e contrastarli giorno per giorno. Noi lo facciamo e vedo che anche oggi lei, Presidente, lo ha ha fatto, come non dubitavamo che avrebbe fatto. Spero che questo avvenga in tutte le istituzioni democratiche, perché sono un bene preziosissimo: non possiamo additarle a ludibrio e usarle magari a scopo televisivo per fare una becera propaganda antidemocratica.

sottolineare i toni e i modi con cui ci si debba rivolgere in quest'Aula, quindi trovo superfluo che da parte nostra si insista nel sottolineare i toni, sicuramente non adeguati del Ministro, o sottolineare le reazioni, a mio avviso, spesso altrettanto non adeguate. Semmai tocca - almeno questo è il mio intento, visto che ho chiesto di parlare sull'ordine dei lavori - sottolineare che siamo ancora in *question time*. L'ordine dei lavori non può essere l'occasione per rinfacciarsi reciprocamente comportamenti o linguaggi sbagliati usati. Questo spetta al Presidente, che lo ha fatto

darsi che fosse assolutamente giusto nei contenuti, ma trovo che sia stato un fuor d'opera da parte del collega Marcucci approfittare di una richiesta di intervenire sull'ordine sull'ordine dei lavori per svolgere un intervento politico. Su questo, Presidente, la prego di registrare il mio intervento.

anche in momenti molto complicati e difficili: la dignità dell'Assemblea, il fatto di invocare il rispetto di quest'Aula e la dignità del Senato della Repubblica.

lei non abbia chiesto scusa a quest'Assemblea. Mi dispiace moltissimo, perché il Presidente l'ha richiamata giustamente, come ha richiamato tutti, ad essere rispettoso ed avere garbo istituzionale, anche quando ci si scontra in posizioni diverse, e io mi aspettavo da lei delle scuse.

Non siamo un circolo ricreativo. Noi abbiamo difeso qui la dignità di quest'Aula, l'abbiamo difesa qui dentro come fuori e non possiamo tollerare, né prima, né tantomeno oggi, che questa dignità sia vilipesa. Noi siamo tutti quanti eletti dai cittadini, caro Ministro, non siamo un circolo ricreativo, non so a cosa lei sia abituato, ma ancora aspettiamo le scuse a quest'Assemblea.